Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 giugno. La seduta di questa mattina si esaurirà nella comunicazione all'Assemblea del calendario dei lavori. Potranno pertanto lavorare le Commissioni, particolarmente quelle impegnate nell'esame del decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. In apertura della seduta pomeridiana di oggi, con inizio alle ore 17, la Presidenza ricorderà la figura del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat nel ventesimo anniversario della scomparsa. Un senatore per Gruppo potrà poi intervenire per 5 minuti. Si passerà quindi alle relazioni sul decreto-legge in materia di sicurezza pubblica. Dopo la discussione e il voto di eventuali questioni incidentali, si aprirà la discussione generale che proseguirà, per concludersi, domani mattina. Sono in corso contatti con il Governo per organizzare - possibilmente nella giornata di domani - un'informativa urgente sui gravi fatti dell'ospedale Santa Rita di Milano. Giovedì pomeriggio è previsto il sindacato ispettivo. La discussione sul decreto-legge in materia di sicurezza pubblica riprenderà martedì 17 giugno, alle ore 11, con le repliche dei relatori e del Governo e 1'inizio delle votazioni sugli emendamenti. Questi ultimi dovranno essere presentati entro le ore 14 di lunedì 16 giugno; i subemendamenti entro le ore 18. Sempre nel corso della prossima settimana, dopo il voto finale sul decreto-legge in materia di sicurezza, si passerà alla trattazione del decreto-legge sul trasporto aereo, che la Camera si accinge a trasmettere in un testo modificato. Ove non concluso in precedenza, tale decreto sarà comunque discusso e votato nella giornata di giovedì 19 giugno, eventualmente anche nel pomeriggio. Pertanto, la prevista seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo. Nuove interrogazioni a risposta immediata saranno poste all'ordine del giorno nel pomeriggio di giovedì 26 giugno.

La seduta è tolta